La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente. Nella seduta di oggi saranno discusse mozioni sulla situazione in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. Dopo l'illustrazione delle mozioni si passerà alla discussione. Alle ore 18 avranno inizio gli ultimi interventi di ciascun Gruppo - per cinque minuti - in discussione. Seguiranno la replica del Ministro degli affari esteri e le dichiarazioni di voto, della durata di cinque minuti per ciascun Gruppo. I disegni di legge istitutivi delle Commissioni parlamentari di inchiesta sull'emergenza SARS-CoV-2 e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, già previsti all'ordine del giorno della seduta odierna, sono rinviati ad altra data. Restano confermati gli altri argomenti previsti in calendario. La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è convocata, per la sua costituzione, giovedì 12 ottobre,

Ha facoltà di parlare il senatore Terzi di Sant'Agata per illustrare la mozione n. 75. Signor Presidente, è un onore poter illustrare i punti fondamentali di questa mozione, presentata dai senatori Malan e Romeo e dalle senatrici Ronzulli e Biancofiore. In questa mozione si prendono si prendono come punto di riferimento le primissime ore di sabato 7 ottobre; quelle ore così drammatiche che abbiamo vissuto davanti allo schermo, con una serie infinita di fotogrammi di terribili scene di violenza; una violenza contro le donne, portate via a forza, e contro i bambini - addirittura ci sono persino dubbi sul fatto che queste foto fossero autentiche - bambini rinchiusi in gabbie e scene terribili di sangue e di uccisioni, che ricordavano episodi come quelli di Breivik a Oslo o del Bataclan o le cose più tremende dello Stato islamico, violenze assolute e assurde dalla nostra umanità nelle sue versioni più degenerate e atroci. Quelle immagini sono nella nostra memoria per sempre; saranno nella memoria dei nostri figli, degli adolescenti o dei piccoli che le hanno guardate e, ancor di più, resteranno nel patrimonio collettivo e nei momenti di disperazione di individui, di parti di un grande popolo, il popolo d'Israele, al quale il il Senato attraverso questa mozione vuole esprimere il suo assoluto e incondizionato sostegno, nonché appoggio *(Applausi)*, solidarietà, comprensione e visione di un futuro che deve essere di pace e sicurezza. Israele ha dichiarato lo stato di guerra; qualcuno ha anche discettato su cosa significasse, se sia stato un passaggio addirittura bellicista nei confronti di Hamas, di un nuovo Stato islamico. È stato sconfitto lo Stato islamico precedente dalla comunità internazionale e ora risorge con forme, modi e una visione millenaristica folle, che è ancora quella di un nuovo Stato islamico, di Hamas, guidato però anche da altri Stati islamici fondamentalisti che probabilmente hanno arricchito di armi micidiali le sue mani

rende coerente con il rispetto del diritto internazionale umanitario quello che sta avvenendo e quello che Israele intenderà fare. È così che deve essere - a mio avviso - interpretata la dichiarazione dello stato di guerra da parte di Israele: entrare cioè in un conflitto sicuramente doloroso, probabilmente lungo

basilari dell'umanità che caratterizzano i nostri popoli e le nostre democrazie anche nelle tragedie delle guerre. Non vi è questione sulle responsabilità di quello che sta avvenendo e che avverrà. Ricade sulla violenza terroristica indiscriminata e folle di un'organizzazione criminale che per la quinta volta, in un crescendo continuo, ha voluto scatenarsi contro un popolo pacifico e sereno,

intessuto dei rapporti importantissimi negli ultimi tre-quattro anni attraverso gli Accordi di Abramo. Tali Accordi sono il fattore di stabilità, di crescita, di comprensione e di amicizia fra i popoli. Gli Accordi di Abramo sono lì. L'Italia dalle missioni che abbiamo visto, dalle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio e dalle missioni già in programma - sono onorato di avere di fronte a me il vice ministro Cirielli,

pace e amicizia, di approccio costruttivo sul piano economico, umano e di sicurezza con i Paesi legati a Israele da accordi regionali. Il Senato, attraverso questa mozione, sottolinea quindi il tema della responsabilità, della condanna e della brutalità dell'aggressione. Sottolinea altresì l'inaccettabilità dei massacri, delle torture e della presa di ostaggi, che deve essere seguita con grande attenzione da parte dell'intera comunità internazionale. L'Italia vuole dare un contributo decisivo nella soluzione, fra le altre, della terribile vicenda di ostaggi presi in così grande numero. numero. Tra l'altro, tutte queste vicende colpiscono anche una ricchissima comunità italiana di doppia nazionalità che risiede a Gerusalemme e in tutto Israele, di cui ha parlato il vice presidente del Consiglio, ministro Tajani, spiegando in dettaglio anche alla Camera l'azione che la Farnesina, il Ministero da lui diretto, sta portando avanti attraverso l'unità di crisi, per mantenere i rapporti in modo capillare per la sicurezza di questi nostri connazionali e la tutela della popolazione civile. Ci sono poi due punti che credo particolarmente rilevanti e sui quali auspico possano essere presi impegni dal Senato in modo consensuale consensuale fra tutte le forze politiche. Il primo impegno è la più ferma condanna a ogni forma di antisemitismo e di richiamo alla definizione di antisemitismo decisa a suo tempo dall'International holocaust remembrance alliance, che include - la cito - il negare agli ebrei il diritto all'autodeterminazione sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele sia un'espressione di razzismo, perché questo è un atteggiamento antisemita: lo è in tutto il mondo e deve esserlo anche in Italia. Dobbiamo prestare particolare attenzione, signor Presidente, a questo aspetto, perché nelle ultime ore, soprattutto ieri, ma ancora oggi, ci sono stati segni che inquietano moltissimo sulla risorgenza di un antisemitismo e di un antistato di Israele, che significa esattamente Come ha spiegato molto bene il premio Nobel Sharansky in alcune manifestazioni su cos'è il nuovo antisemitismo, non ci si può in alcun modo mascherare attorno ai distinguo sull'opposizione a cosa fa o meno lo Stato di Israele per indicare poi espressamente che - e qui cito un alto funzionario delle Nazioni Unite, che in un recente convegno ha avuto l'ardire di asserirlo - in realtà il problema dei diritti umani in Palestina è irrisolvibile finché ci sarà lo Stato di Israele. Ecco, questo è l'antisemitismo che deve essere condannato e sul quale deve essere sostenuto un grande sforzo

la commissione presieduta dalla senatrice Liliana Segre e questo impegno deve essere portato avanti, perché l'antisemitismo ufficiale, proclamato e conclamato dalla Carta di Al-Fatah - che precisa al primo punto che lo Stato di Israele non deve esistere - dalla Carta di Hamas, dalla Carta di Hezbollah e dalle dichiarazioni dello Stato islamico iraniano fa parte di una propaganda antisemita a livello globale. Queste nuove forme di antisemitismo devono essere combattute. La seconda questione importante e conclusiva sono i finanziamenti ad Hamas, organizzazione terroristica con componenti mafiose, come tipo di gestione. Non c'è *governance* in quel mondo, per cui non è immaginabile che finanziamenti ad Hamas possano avere anche solo la parvenza di essere destinati a persone in stato di necessità, individuate dalle entità donatrici o dalle organizzazioni internazionali o dagli Stati e dalle persone in buona fede che effettuano le donazioni con organizzazioni non governative.

tutto l'arco costituzionale di Camera e Senato riuscisse a lavorare per un testo unitario. E se ciò non è stato possibile, è perché c'è stata una fuga in avanti dei partiti di maggioranza, che hanno annunciato già da sabato la presentazione di una mozione qui in Senato, rendendo quasi superfluo il ruolo delle opposizioni, che invece in questo frangente potevano dare un contributo per un'unità auspicabile in un momento così drammatico.

in Israele e le successive azioni che Israele, per la propria autodifesa, ha compiuto nella striscia di Gaza. Si parla per lo più di vittime civili e credo che non si possa prescindere da due elementi, entrambi centrali. Il primo elemento è una ferma, decisa condanna di ciò che è accaduto nelle prime ore di sabato mattina, la cui responsabilità è attribuibile esclusivamente a Hamas, gruppo terroristico riconosciuto come tale, oltre che in Europa, in tanti Paesi del mondo. La seconda considerazione, però, imprescindibile in qualsiasi testo, è che debbano cessare le morti civili, che siano palestinesi, israeliane o di qualsiasi altra nazionalità.

e arrivare a una situazione che consenta a chi sta in quelle terre di fuggire, ove possibile, con la creazione di corridoi umanitari. È sostanzialmente questo il centro dell'impegno che noi chiediamo al Governo, e cioè che si adoperi

nel chiedere un immediato cessate il fuoco; nel chiedere che nella risposta - come certamente sarà, anche se alcune dichiarazioni portano a pensare con preoccupazione al prossimo futuro - ci si muova sempre all'interno del diritto internazionale. La creazione dei corridoi umanitari si inserisce in questo contesto di diritto internazionale, così come la preghiera che tutti noi facciamo, ovvero che non ci siano più civili che cadono sotto le bombe degli uni e degli altri.

del Governo, colleghi, l'attacco brutale e indiscriminato che Hamas ha condotto nelle scorse ore nei confronti di Israele, della sua popolazione inerme, della sua realtà territoriale impone correttamente e giustamente una modifica all'organizzazione dei nostri lavori. Siamo quindi dell'opinione che sia stato giusto modificare il nostro modo di lavorare e spostare ad altra data le determinazioni che dovevamo assumere. La questione che oggi ci si pone di fronte è di grande ed estrema gravità e solo una miopia potrebbe immaginare che non ci coinvolga, non ci tocchi, non sia qualcosa che parla anche alla nostra realtà nazionale. E questo non solo perché in generale, ogni volta che il diritto internazionale viene denegato dall'impiego di armi che colpiscono le popolazioni civili, un Parlamento di una Repubblica democratica come

Già questo basterebbe di per sé per giustificare il lavoro che stiamo compiendo e che - lo preannuncio vogliamo fare in modo che non venga interpretato come un'occasione perduta. Naturalmente ogni forza politica, ogni Gruppo parlamentare, con le proprie sensibilità e le proprie peculiarità, legge questa vicenda, che è una delle più controverse della storia, con la propria lente d'ingrandimento. Noi non vediamo con preoccupazione la polifonia delle discussioni, anzi questo è il sale della democrazia, è l'elemento che ci caratterizza. Noi riteniamo però, partendo da queste diversità e angolature differenti, ci possano anche essere dei momenti di coesione che leghino anche le forze politiche più diverse fra loro in quest'Aula all'interno della salvaguardia di alcuni valori fondamentali. Riteniamo inoltre che si possa anche tradurre in una possibile espressione di un ordine del giorno che, indipendentemente dal voto delle singole mozioni, possa trovare un suo punto di coesione e di caduta che tenga insieme il più possibile l'espressione unitaria di questo Parlamento. solo della questione che riguarda un aspetto di carattere generale, perché quello che è accaduto nelle scorse ore in Israele non è solo

Quei ragazzi massacrati in quel deserto, in quel Bataclan israeliano, ci parlano, ci interrogano e chiedono che la nostra voce non sia silente. Per questo è giusto che oggi noi esprimiamo una nostra una nostra posizione. Per il nostro Gruppo interverranno nel merito i senatori Calenda e Renzi, per cui non anticipo le espressioni di merito che i colleghi faranno successivamente, se non per un aspetto, signor Presidente, e cioè il fatto che noi dobbiamo riflettere sui motivi di quello che sta accadendo. Far politica, infatti, non è la declamazione di generici valori e non è neanche il racconto di ciò che sta accadendo: far politica è l'analisi e la comprensione di un fatto storico, la capacità di intervenire per modificarne le determinazioni. Non possiamo quindi non vedere che l'attacco di Hamas è stato lanciato nel momento in cui Israele e Arabia Saudita stavano immaginando di estendere a quel sistema di relazioni internazionali il cosiddetto Patto di Abramo, che già negli scorsi anni ha visto una intesa tra gli Emirati Arabi Uniti, il Marocco e Israele. È altrettanto evidente che dietro questa operazione c'è il duplice tentativo, all'interno del composito mondo musulmano, con la presenza dell'Iran, di creare condizioni di difficoltà nei confronti dell'Arabia Saudita e, più in generale, all'interno del Medio Oriente, di creare condizioni di destabilizzazione di un teatro, quello del Mediterraneo, nel quale proviamo a guardarci attorno, cari colleghi, a proposito del fatto che questo è un attacco ai valori e al sistema occidentale. Prendiamo un compasso, puntiamolo attorno a quel lago che è il Mediterraneo e guardiamo tutti i *flash point* che vengono accesi, che sono stati accesi e si stanno accendendo: vi è la drammatica spirale dell'Ucraina, su cui abbiamo per lungo tempo discusso; le vicende terribili del Nagorno-Karabakh e degli oltre 100.000 armeni costretti a scappare mentre venivano distrutte le loro realtà identitarie (la distruzione delle croci e delle chiese). sono le vicende mai sopite e sempre complesse dei curdi e ora il Medio Oriente che si riaccende ancora. Se continuiamo a usare il compasso, arriviamo al Nord Africa e alla situazione molto complessa dell'Egitto, che potrebbe trovare un'ulteriore compressione dall'ondata migratoria che sta per partire dalla striscia di Gaza; oggi è stato chiuso il valico di migrazione e di scambio fra Gaza e l'Egitto. Per non parlare della drammatica vicenda dei Balcani occidentali, dove nelle scorse settimane il posizionamento di truppe serbe, che che possiamo dire filo-russe, ai confini del Kosovo, ha nuovamente alzato il livello della tensione. Sono teatri nei quali - penso al Kosovo e al Libano - i nostri militari stanno svolgendo forze di interposizione di pace nell'ambito di missioni internazionali. Ora capite che tutto si tiene e che l'innesco di un elemento di complessità, o peggio ancora un elemento di guerra, rischia di scatenare teatri che inevitabilmente comportano il coinvolgimento del nostro Paese. se anche fossimo miopi e guardassimo da un'altra parte - e non lo vogliamo e non lo dobbiamo fare - la storia si incaricherebbe molto presto di risvegliarci e di richiamarci rispetto ad un tema. Concludo, signora Presidente: si discute molto del tema dei valori. Ebbene, bisogna che noi declamiamo con grande forza che Israele è una democrazia e che Hamas è un sistema militare terroristico che vuole denegare i valori fondamentali di quella democrazia. E vorrei dire a coloro i quali guardano con una certa sufficienza e leggerezza ai fatti di queste ore di venire a guardare come le democrazie affrontano i problemi: i problemi si discutono nei Parlamenti, nelle Aule, nella democrazia. Quando si prende in mano un kalashnikov, quando si lancia un missile su popolazioni inermi, quando si utilizza lo strumento della guerra per colpire un proprio interlocutore, immediatamente la situazione diventa inaccettabile. È anche per questo, per la difesa di questi valori e modelli, noi riteniamo sia giusto che oggi il Parlamento italiano si esprima, perché - come ha detto qualcuno la peggiore delle democrazie è sempre migliore della migliore delle dittature.

di quest'Assemblea il saluto e il ringraziamento del Presidente della Knesset, che ho sentito telefonicamente e a cui mi sono permesso di formulare la solidarietà di tutti quanti

cordoglio alle vittime che da sabato scorso scolpiscono una delle

dopo questa discussione generale, organizzata - devo dirlo - con l'impegno di tutte le forze politiche un po' all'ultimo momento, per le ragioni che proverò a ricordare a tutti noi e che devono responsabilizzarci, in momenti come questo, a ricercare sempre e comunque l'unità della Repubblica. Signor vice presidente Tajani,

di sottolineare qui all'attenzione dell'Assemblea alcune riflessioni legate al tentativo che tutti i partiti di opposizione - che mi permetto di interpretare - hanno fatto già da sabato pomeriggio: l'Aula del Senato era chiusa, ma tra noi è partito immediatamente un tentativo di costruirvi, signor Presidente, un momento di confronto con un unico obiettivo,

signor vice presidente del Consiglio, devo confessarglielo: non abbiamo capito fino in fondo perché la maggioranza

al Senato della Repubblica come alla Camera dei deputati, di partire da un documento che i 27 Paesi dell'Unione europea avevano adottato. dice chiaramente che l'Unione europea condanna con la massima fermezza gli attacchi multipli e indiscriminati da parte di Hamas e tutta Israele deplora profondamente la perdita di vite umane, ribadendo che l'Unione europea chiedeva, come chiede, la cessazione immediata degli attacchi e delle violenze insensate che non faranno altro che aumentare le tensioni sul terreno e compromettere le aspirazioni di pace del popolo palestinese, che non è Hamas. che non è Hamas. Ripeto: il popolo palestinese non è Hamas e quando si dice, come si è detto, che "due popoli,

nel nostro recente passato non hanno funzionato. Non vorrei che ripartissimo dagli errori che abbiamo alle spalle. Il tema è tutto qua, signor Vice Presidente del Consiglio. Noi ci auguriamo che quella posizione assunta dai 27 Paesi dell'Unione europea diventi la posizione... La prego di concludere perché siamo d'accordo nel rispettare i tempi.

quando diceva: «Ho sempre pensato che la maggioranza del nostro popolo vuole la pace ed è pronta ad assumersi dei rischi in nome della pace». Ebbene, in questo momento sia il popolo israeliano che il popolo palestinese vivono continuamente dei rischi in cambio della guerra. Noi questo non possiamo accettarlo e dobbiamo fare di tutto per far sì che tutto questo finisca.

Egregio Presidente, onorevoli colleghi, Vice Presidente del Consiglio, vorrei associarmi a quanto detto dal senatore Patuanelli. Ovviamente la nostra mozione parte da un dato di condanna senza se e senza ma rispetto a quanto avvenuto, in quanto gli atti terroristici non ci appartengono. Tengo sempre a sottolineare, essendo un uomo del Novecento, che ho combattuto ovviamente anche il terrorismo nero e rosso,

non la guerra. Anche oggi in questa sede, di fronte a un fatto drammatico come questo, credo che noi dobbiamo porre il problema

affrontare la situazione per come è. Dobbiamo sapere che in questi anni, in questi ultimi anni, il popolo palestinese è stato sostanzialmente sempre marginalizzato, respinto e nello stesso tempo è stata fatta un'azione di

Tajani, colleghi, è fondamentale che oggi da quest'Aula arrivi un messaggio forte e unitario a sostegno di Israele per il vile attacco terroristico subito. È fondamentale in quanto giusto, ma è ancor più fondamentale perché è già partito un assordante rumore che ha l'obiettivo di confondere l'opinione pubblica. Sentiremo dire che la situazione è talmente complessa da non poter scorgere i torti e le ragioni; che le responsabilità sono del Governo israeliano, dell'Occidente, degli USA e via dicendo. Qualcuno spiegherà - e per la verità è già accaduto - che è stato assurdo organizzare una festa vicino ai confini di Gaza, come se questo rappresentasse una variabile di una qualche rilevanza rispetto a quanto accaduto. Qui il nocciolo della questione è che una democrazia liberale, amica dell'Italia e dell'Europa, è stata attaccata da un gruppo di terroristi senza scrupoli, che hanno ucciso e sequestrato civili inermi. Noi stiamo con Israele, senza se e senza ma. Questo va detto in modo chiaro e netto perché si ripeterà nei *talk show*, sulla stampa e sui *social* ciò che è accaduto alla vigilia dell'invasione russa e che purtroppo continua ad accadere quotidianamente: dosi massicce di disinformazione faranno breccia in un'opinione pubblica comprensibilmente stanca di dover prendere posizione su conflitti che appaiono lontani e che invece sono vicinissimi. Il terrorismo non è mai lontano. La sua diffusione mette a rischio l'Italia e gli altri Paesi europei, come i nostri amici francesi sanno molto bene. Si cercherà ogni scappatoia pur di non assumerci le responsabilità che competono ad una democrazia liberale, che ha l'obbligo morale e l'interesse nazionale di andare in soccorso di un'altra grande democrazia liberale, sorella dell'Italia, dell'Europa e dei Paesi occidentali. Ci sarà nuovamente l'uso della parola «pace» per assolvere gli aggressori e ci saranno partiti e movimenti politici che cercheranno, così come accade per la guerra ucraina, di usare la stanchezza della popolazione per cercare di raccattare qualche consenso. Noi saremo sul fronte opposto. Per una generazione cresciuta nel tempo della fine della storia risvegliarsi in un'epoca di ferro è difficile. La tentazione di girarsi dall'altra parte è grande e persino comprensibile, ma non sarà possibile. La storia è tornata alle porte dell'Occidente dell'Europa il nostro compito è persuadere i cittadini italiani che non c'è alternativa a quella di assumerci per intero la responsabilità che deriva da questo fatto. Parliamo, appunto, di fatti: Hamas è un'organizzazione terroristica; il braccio militare di Hezbollah è un'organizzazione terroristica; la Siria è uno Stato canaglia, così come l'Iran e la Russia, che di questi Paesi è un alleato prezioso. Il ruolo della Russia in Medio Oriente, dalla guerra siriana in poi, è andato crescendo, con il chiaro obiettivo di destabilizzare l'area e danneggiare gli Stati alleati dell'Occidente. Troppo spesso ci siamo limitati ad osservare senza intervenire e i risultati sono quelli che vediamo: un mondo in fiamme e la nostra sicurezza compromessa. Anche la tempistica di quanto accaduto lascia immaginare una mano straniera interessata non solo a a interrompere il dialogo tra Israele e Arabia Saudita, ma anche a fiaccare l'Occidente rispetto all'impegno sul fronte ucraino. Si va dunque delineando un asse di nemici dell'Occidente alle nostre porte, un asse rispetto al quale dobbiamo assumere una postura dura. La presa di potere di Hamas nella striscia di Gaza ha determinato una condizione di oggettiva impossibilità di dialogo. La risposta dell'Unione europea deve essere compatta, come quella messa in atto rispetto all'invasione russa dell'Ucraina. Cari colleghi, ci sono mille morti israeliani, di cui 200 civili e più di 100 persone sequestrate e minacciate di morte: questo in primo luogo è ciò che conta. Hamas ha iniziato un conflitto nella maniera più vigliacca e inumana possibile: le conseguenze di questo atto criminale non possono essere fatte ricadere su Israele. Tutti ci auguriamo che questo conflitto duri un tempo limitato e che la diplomazia possa avere un ruolo, ma dobbiamo essere consapevoli che ciò non sarà possibile prima della definitiva sconfitta militare di Hamas. Risparmiamoci la retorica delle buone intenzioni: non serve a noi e non serve al Medio Oriente. Diamo un messaggio chiaro: oggi qui siamo tutti israeliani.

solidarietà al popolo d'Israele, perché Israele - ogni volta lo ribadiamo - è l'unica democrazia che c'è in quel lembo di terra, dove il resto degli Stati - qualcuno ha definito poco fa la Siria uno Stato canaglia - ha una diversa situazione. Israele è l'unico Paese dove si svolgono le elezioni. Anzi, ripetutamente, perché Israele - come sappiamo - negli ultimi anni ha faticato nella Knesset a trovare una maggioranza e quindi ha votato con una frequenza enorme. È anche un lembo di Occidente, per tradizione di vita, per cultura, per provenienza di tante persone da una diaspora mondiale, figlia delle persecuzioni che gli ebrei hanno subito, ed è una realtà a noi vicina; anzi, molte volte si è addirittura sostenuto - lo diceva anche il presidente Berlusconi talvolta - che Israele dovesse entrare nell'Unione europea. C'è quindi una vicinanza per ragioni storiche e morali. C'è poi la storia delle persecuzioni che gli ebrei hanno subito, non solo con l'orrore dell'Olocausto del Novecento, ma nel corso dei millenni e della storia. È un popolo assediato, un popolo perseguitato. Vedo ancora in queste ore ricominciare dei distinguo: c'è la reazione in corso? Beh sì, Israele ha dichiarato uno stato di guerra, sta nascendo un Governo con tutte le componenti politiche che superano le divisioni di fronte a quella che è stata un'esplosione di odio e di fanatismo, anche con elementi di fondamentalismo religioso, perché avrete visto anche voi, come me, nelle immagini urlare «Allah *Akbar*» da parte di molti di questi invasati di Hamas. Devo anche dire che nel mondo palestinese non solo Hamas, ma tante organizzazioni anche ufficiali nei loro statuti e principi fondamentali hanno sempre proclamato la necessità di cancellare Israele. Quindi, giustificazionismo rispetto a condizioni difficili. Non c'è dubbio, Gaza è un luogo con mille problemi, è una realtà che certamente alimenta odi e rancori. Però forse bisognerebbe tornare indietro con la storia

di questi giorni. Le immagini di questa strage sono state orripilanti. Purtroppo in quella parte del mondo le guerre sono state frequenti in tutta la fase del Dopoguerra

e raccontava la tragedia perenne che si rinnova nella sinagoga di Roma e in una dimensione ovviamente molto più gigantesca in Israele, nelle guerre, negli stillicidi, negli attentati, nel soldato che l'altro giorno in Egitto impazzisce e ammazza

palestinese *(Applausi)* non possono essere più tollerate. Anche in queste ore a me pare assurdo che ci debbano essere - a Roma forse no, ma a Milano - due manifestazioni; anche il sindaco Sala - l'ho letto su un'agenzia ha detto di non venire sotto il Comune, come se fosse un dibattito di una trasmissione televisiva, con quelli a favore e quelli contro. Non esiste l'equidistanza rispetto a queste vicende *(Applausi)*, quindi ribadisco senza nessuna enfasi retorica la nostra posizione contro il fondamentalismo, contro il terrorismo, contro Hamas e contro coloro che devono cancellare da ogni atto giuridico e politico del mondo palestinese la distruzione di Israele, atto che noi non consentiremo. Vogliamo tutti la *de-escalation*, come ha invocato anche

a giovani inermi. Voglio subito sgombrare il campo da possibili fraintendimenti: il MoVimento 5 Stelle esprime l'assoluta e ferma condanna a questo infame atto di violenza e terrorismo contro il popolo di Israele; è un crimine che non ha alcuna giustificazione. Come ho già detto più volte in quest'Aula ripetendo parole non mie, la violenza genera violenza e non è mai la risposta. Presidente del Consiglio, noi pensiamo che il Governo italiano che lei qui rappresenta debba rivolgere un appello a Israele perché eserciti il suo legittimo diritto di difesa nel rispetto del diritto umanitario internazionale e che la risposta non sia una punizione collettiva indiscriminata. Capiamo benissimo che la sete di vendetta o il "dente per dente" siano le reazioni che prima di tutte possano apparire più giuste a fronte di atrocità subite. Operando così, però, si alimenta odio per molte generazioni; reagire tagliando luce, acqua e gas alla popolazione palestinese è un atto che colpisce soprattutto i civili, quelli che il conflitto lo subiscono senza volerlo, non un legittimo diritto di difesa contro obiettivi militari. Ricordo che tagliare le forniture di servizi vitali come luce, acqua e gas è una pratica di assedio condannata dall'ONU, come ribadito dall'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk. Riteniamo, signor Ministro, che si debba agire per chiedere e ottenere l'immediata apertura di corridoi umanitari, per consentire l'evacuazione temporanea di bambini, donne e anziani dalla striscia di Gaza e, come richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità, per consentire di raggiungere i civili di Gaza con forniture mediche essenziali. Al tempo stesso, è urgente che si operi in ogni sede e con ogni mezzo diplomatico per far liberare gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. So che il suo è un compito arduo, signor Ministro: lo sarà. È importante, ministro Tajani, impegnarsi a lavorare al fine di evitare che il conflitto produca ulteriori massacri e che si allarghi ai Paesi vicini. Mi riferisco *in primis*, ovviamente, al Libano, dove gli Hezbollah potrebbero effettuare un attacco ad Israele, impegnato com'è attualmente nella risposta militare ad Hamas. Sappiamo tutti che qualche razzo, qualche missile, è già stato sparato dal Nord e che è in corso una risposta di Israele anche in quel territorio. Ricordo che ci sono oltre mille nostri militari. È già stato detto, ma è meglio ribadirlo: ci sono mille nostri militari che fanno parte della missione UNIFIL, nei Caschi Blu dell'ONU. L'obiettivo dovrebbe essere quello di rimettere al centro del dibattito la soluzione politica dei "due popoli, due Stati". Lei deve coinvolgere i suoi omologhi europei e ritengo che questa sia un'assoluta priorità, per l'Europa tutta e anche per il mondo intero. Ammettiamolo: la disattenzione della comunità internazionale verso la questione israelo-palestinese ha di fatto interrotto il difficile processo di pace che si era avviato. Poi è arrivata anche la proposta di Trump, che prevedeva di fatto lo smembramento totale della Palestina e la perdita di Gerusalemme come città condivisa, facendola diventare la capitale di Israele. Questa proposta è stata, a parer mio, una umiliazione per le aspirazioni del popolo palestinese, che, in contemporanea, si è trovato anche abbandonato dai suoi storici sostenitori del mondo arabo. Il riavvicinamento a Israele degli Emirati, del Bahrein e anche dell'Arabia Saudita non ha fatto altro che isolare i palestinesi. Se guardiamo l'attuale situazione mondiale, possiamo notare che il conflitto israelo-palestinese è parte integrante di un'instabilità globale, che deriva, sì, dal prolungarsi del conflitto in Ucraina, ma anche da una destabilizzazione globale che va dall'Europa ai Balcani fino al Caucaso. Pensiamo ad esempio al conflitto in Armenia con l'Azerbaijan, al Maghreb, alla Libia al Sahel in Niger. Sono oltre sessanta i Paesi in conflitto nel mondo. C'è da augurarsi che questo conflitto non ne scateni altri. Signor Ministro, noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per fermare diplomaticamente questo e gli altri conflitti. Sono convinto che nessuno in quest'Aula sia a favore di qualsivoglia guerra. Dobbiamo, sì, denunciare le barbarie dei gruppi terroristici, ma anche avere il coraggio di evidenziare gli effetti, a volte catastrofici, delle politiche di Governi amici.

che da subito, senza tentennamenti e senza indugi, si è immediatamente schierato a fianco di Israele e del popolo israeliano, condannando senza se e senza ma il vile attacco contro Israele compiuto da un'organizzazione terroristica palestinese. colleghi, organizzazione terroristica, perché le parole sono importanti ed è necessario chiamarli con il loro vero nome: sono dei terroristi, delle belve disumane, che hanno rapito, violentato e ucciso una ragazza, portandola in giro nuda come un trofeo. Hanno sparato a bambini innocenti, hanno rapito donne anziane, decapitato soldati israeliani, massacrato famiglie e distrutto scuole, asili, ospizi: veri e propri crimini contro l'umanità. Hamas e la *jihad* islamica hanno dimostrato per l'ennesima volta il loro vero volto, quello di un brutale fondamentalismo che non fa sconti a nessuno, con buona pace tra l'altro di una certa sinistra, che tanta fatica fa a pronunciare nella stessa frase Hamas e terrorismo, o dei centri sociali, che in alcune scuole inneggiavano ad Hamas e cantavano "che bello quando brucia Tel Aviv". A tal proposito, vorrei ringraziare il ministro Valditara per aver avviato delle ispezioni. poi a chi strizzava l'occhio all'Iran, grande sostenitore del fondamentalismo palestinese e Paese con il quale è necessario essere intransigenti e fare di tutto per evitare che possa diventare una potenza militare nucleare; l'arma nucleare in mano in mano agli *ayatollah* creerebbe ancora più instabilità, violenza e devastazione di quella attuale. Nutro tra l'altro, Ministro, profonda tristezza e sconcerto nel vedere che anche in città europee vi sono scene di giubilo da parte di qualcuno che, con la bandiera palestinese al collo, festeggia l'uccisione di innocenti israeliani, soprattutto civili. Vorrei ricordare che, qualche giorno prima dell'attacco, Hezbollah, milizia libanese filo-iraniana e grande alleata proprio di Hamas, annunciava la sua intenzione di rilasciare centinaia di migliaia di migranti presenti in Libano per indirizzarli verso l'Italia e l'Europa, al fine di destabilizzare il nostro Paese e il nostro continente, ribadendo quello che noi della Lega abbiamo già denunciato da tempo: l'uso dei migranti come arma ibrida. E proprio quando è in corso questa macelleria islamista in Israele, c'è ancora qualcuno che vorrebbe aprire le porte a chi ci è ostile e che non vede l'ora di cambiare la nostra cultura, il nostro modo di vivere e il nostro modo di pensare. Quello che sta succedendo succedendo non è solo una guerra tra israeliani o palestinesi: siamo tutti noi occidentali ed è la nostra seppur imperfetta civiltà ad essere messa nel mirino del fanatismo e del terrorismo islamico. È necessario allora essere estremamente chiari: non bisogna cercare giustificazioni pretestuose per questi terroristi, basta con i "ma Israele", "per il governo di Israele", "però noi occidentali". Bisogna iniziare a pensare in modo diverso e a trattare questi assassini in maniera assolutamente adeguata. È il momento di condannare queste belve e di schierarsi. Come Italia non possiamo avere dubbi: fermare subito tutto il supporto a Hamas e alle associazioni che intrattengono rapporti con questa organizzazione islamista, onde evitare che finanziamenti italiani ed europei finiscano in mano ai terroristi e ai loro fiancheggiatori. *(Applausi)*. e supporto incondizionato alle istituzioni israeliane e al suo popolo. Spingere per un'azione diplomatica, ove possibile, volta al rafforzamento degli Accordi di Abramo, per un coinvolgimento nel processo di pace e stabilizzazione anche dell'Arabia Saudita, per isolare Hamas e i suoi sostenitori. Permettetemi infine un pensiero, in queste ore di apprensione, alle Forze armate italiane presenti nell'area, dai Carabinieri a Gerico ai militari che operano nel contingente UNIFIL nel sud del Libano. *(Applausi)*. Un grazie a queste ragazze e a questi ragazzi, che mantengono alto il tricolore anche in queste occasioni. Gerusalemme rappresenta il baluardo dei valori occidentali nel Medio Oriente. Israele lotta per la sua esistenza, per esistere libera e democratica, contro il terrorismo islamico di Hamas e dei fondamentalisti jihadisti, che la vogliono annientare. Per questo ribadiamo con certezza e convinzione: viva la democrazia, viva la libertà, viva l'Occidente, viva Israele!

ha detto giustamente il senatore Boccia che, come per l'Ucraina, anche la drammatica vicenda dell'aggressione di Hamas allo Stato di Israele ci dà l'occasione per dimostrare il valore dell'unità tra le forze parlamentari in frangenti di questo tipo. Mi auguro che il dibattito qui al Senato si concluda con un voto un voto unico ed unanime, perché coltivare il comune sentire significa una cosa molto importante: riporre nel cassetto la faziosità. Colleghi, la faziosità o gli *slogan*, anche in questo dibattito, non aiutano a capire questioni complesse e soprattutto non aiutano a portare a intelligenti soluzioni. Oggi, in questo Senato, siamo tutti, dal primo all'ultimo, israeliani senza se e senza ma. Abbracciamo idealmente la comunità ebraica del nostro Paese che oggi è in trepidazione, peraltro nel 41° anniversario dell'attacco alla Sinagoga di Roma e della morte del piccolo Stefano. Non ci sono parole per definire la bestialità e la barbarie contro civili inermi, 40 bambini uccisi e decapitati in un *kibbutz*. Tanti bambini però in questi giorni muoiono anche dall'altra parte e sono sempre bambini. In astratto, anche la causa teoricamente più nobile non potrà essere mai portata avanti con metodi disumani. Ecco dunque che noi dobbiamo riflettere sull'obiettivo di Hamas in questi giorni. Per noi è evidente: bloccare la normalizzazione di rapporti tra Israele e i Paesi sunniti dell'area, in particolare l'Arabia Saudita. Gli Accordi di Abramo sono l'obiettivo e il timore. Dietro Hamas si staglia netto il profilo della principale potenza sciita di quell'area che, pur dichiarandosi non responsabile, ha già espresso ogni possibile solidarietà ad Hamas. Iran, Hamas e naturalmente il braccio armato degli Hezbollah dal fronte siriano libanese contribuiscono alla tenaglia che mette alla corda uno Stato democratico come quello di Israele. Altro obiettivo è quello di destabilizzare i Paesi arabi moderati e l'operazione - attenzione perché questo è il punto - avviene utilizzando spregiudicatamente la questione palestinese che è tutta altra cosa e che non può essere in alcun modo non ho udito altri in questo dibattito, ma io credo che noi dobbiamo fare anche un esame di coscienza. Noi, come Europa e come Italia, abbiamo grandissime responsabilità nell'aver rimosso dall'agenda multilaterale delle politiche internazionali la questione israelo-palestinese. Questo è stato il più grande regalo agli estremisti di Hamas, che oggi si propongono come l'unica soluzione per la disperazione di un popolo. È ovviamente una mistificazione; lo capiamo tutti che questa è una mistificazione perché i primi a soffrire le conseguenze di questa azione disumana saranno proprio i palestinesi, le migliaia di uomini e donne a cui non possiamo vietare di sostenere quello che la politica italiana ha sempre sostenuto; dagli Accordi di Oslo del 1993 in poi abbiamo sempre sostenuto, come anche questo Governo giustamente "due popoli, due Stati". No dunque all'identificazione inaccettabile tra le bandiere verdi di Hamas e quelle dello Stato palestinese. Ovviamente qualcuno oggi ritiene irrealistico parlare in futuro della possibilità che ci sia uno Stato palestinese. Colleghi, se questo avverrà, aggiungerà un errore drammatico agli orrori di questi giorni. Noi dobbiamo assolutamente tenere ferma la barra anche in un momento di questo tipo. Dobbiamo lavorare perché la comunità internazionale capisca che un popolo non può non avere una sua prospettiva e ovviamente avere ben chiaro che Hamas è fuori da questo circuito, è un gruppo terroristico che non può avere alcuna indulgenza da parte della comunità internazionale e che oggi è il vero nemico della causa palestinese. Infine - e ho terminato, Presidente - non ho espresso alcun giudizio sulla politica attuale del Governo d'Israele. I Governi passano, i Paesi rimangono e io spero che anche in questo caso si confermi la tradizione.

non avevo memoria, va condannato. Il Gruppo Fratelli d'Italia, come ha già fatto chi mi ha preceduto, ovviamente esprime la massima, totale, incondizionata e incondizionabile solidarietà al popolo israeliano.

disarmatiti all'interno di un territorio sovrano, che, come tale, non può quindi che essere fortemente condannato, senza alcun tipo di perplessità. Non è questo il momento dei distinguo e non è oggi il momento delle valutazioni storiche o delle evoluzioni, su cui, per carità, possiamo fare tutte le riflessioni del mondo,

allora che oggi abbiamo il compito di raccontare fuori da qui quello che sta accadendo, perché siamo circondati - anche questo è già stato detto, ma è vero - da conflitti sempre più numerosi, che sembrano lontani, ma che hanno ricadute reali sulla nostra sicurezza, sulle nostre prospettive di sviluppo anche economico e sulla capacità italiana e occidentale di difendere i nostri valori, il nostro stile di vita e i nostri credo. Se sul fronte est abbiamo la vicenda russo-ucraina, la vicenda armena-azera e la vicenda serbo-kosovara e oggi si alimenta anche in un'altra regione con uno scenario sempre più instabile un qualcosa di così drammaticamente pericoloso, è chiaro che serve l'attenzione di tutti noi e ovviamente del Governo per far sì che sia l'Europa la protagonista di un Mediterraneo che ne fa parte e

perché è legittima difesa e questo non si può assolutamente mettere in discussione, ma dovremmo anche porci il problema del domani. È quindi evidente che oggi dobbiamo fermarci alla solidarietà piena e assoluta al popolo israeliano e, da domani, riuscire a costruire attraverso il... finestra"). Prima di dare la parola al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, Grazie,

dal mio intervento alla Camera stamattina ad ora e rispondere a qualcuna delle osservazioni che gli oratori hanno fatto nel corso di questo dibattito. Sono reduce dalla riunione virtuale dei Ministri degli esteri dell'Unione europea dedicata alla crisi in atto. Vi è collaborazione con I due Ministri degli esteri di Israele e Palestina non hanno ritenuto, nelle attuali circostanze, di partecipare alla riunione alla quale erano stati invitati, oggi, dall'alto rappresentante Borrell questo è un ulteriore segnale della difficoltà della situazione. Nel corso della riunione, ho riaffermato la solidarietà a Israele e la forte condanna delle azioni terroristiche perpetrate da Hamas, oltre che l'appello per il rilascio immediato degli ostaggi, a cominciare da anziani, donne e bambini. Ho ribadito l'impegno del Governo italiano per prevenire ogni possibile allargamento del conflitto sul piano regionale, con particolare riferimento al confine con il Libano e attraverso un coinvolgimento attivo dei Paesi arabi più interessati. Ho riferito anche sulla mia imminente missione in Egitto che si svolgerà domani. Durante questa missione incontrerò il *leader* della Lega araba, incontrerò il presidente al-Sisi e il Ministro degli esteri dell'Egitto per affrontare con questi *leader* la situazione in atto e anche per cercare di far sì che non ci sia una crasi con il mondo arabo che vuole il dialogo, che vuole il confronto, che ha anche un dialogo con Hamas e con il mondo palestinese al fine, in questo momento, di cercare di avere eventuali corridoi umanitari per salvare gli ostaggi, tra i quali probabilmente ci sono anche due cittadini italiani che hanno il passaporto italiano, ma anche quello israeliano. Non abbiamo notizie ulteriori su di loro: mancano all'appello, il figlio li sta cercando, ma probabilmente sono fra gli ostaggi che sono nella striscia di Gaza. Continueremo a fare di tutto per cercarli e per liberarli. liberarli. Durante la riunione dei Ministri degli esteri sono stati anche chiariti i termini dell'annunciata revisione dell'ingente pacchetto di aiuti ai palestinesi, che ha lo scopo di evitare che anche per vie indirette parte dei fondi possa pervenire ad Hamas. Resta ferma la determinazione dell'Unione europea ad aiutare il popolo palestinese, che va tenuto distinto dall'organizzazione terroristica. Ho sottolineato in maniera ferma l'importanza di vigilare in maniera attenta e severa la gestione e gli effettivi destinatari dei fondi europei, anche quelli della cooperazione: non devono finire non solo nelle mani dei terroristi, ma neanche nelle mani di coloro che utilizzano questi fondi per fare propaganda antiebraica e razzista. Stiamo facendo lo stesso, come ho sottolineato oggi alla Camera e lo ribadisco in quest'Aula, con i fondi italiani della cooperazione. In questa sede non posso fare altro che ribadire la posizione

Quello che abbiamo visto, soprattutto contro la popolazione civile, è inaccettabile; il modo con il quale sono trattati gli ostaggi è inaccettabile. Profanare i morti, anche se nemici, è inaccettabile. Il vilipendio dei cadaveri è una cosa vergognosa: è da vili, non da combattenti, perché nessun combattente ha il diritto di profanare il nemico caduto. Purtroppo ci sono molti morti, molti feriti: gli israeliani certamente sono stati i primi, penso ai ragazzi innocenti uccisi durante un *rave,* ostaggi, ai bambini piccolissimi: circolano immagini raccapriccianti sulla detenzione di questi bambini. Ci sono vittime tra la popolazione palestinese, oltre che naturalmente tra i terroristi di Hamas. di Hamas. Onorevoli senatori, vorrei anche aggiornarvi sulla situazione degli italiani che sono in Israele. Come sapete, sono circa 18.000 i cittadini italiani residenti in quel Paese, quali hanno il doppio passaporto; fra questi ci sono circa 1.000 giovani italiani che hanno anche passaporto israeliano, che stanno svolgendo il servizio di leva nell'esercito israeliano.

che erano e sono in Israele per motivi di lavoro, di viaggio, molti sono pellegrini. Desidero ringraziare ancora una volta tutti i funzionari dell'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, tutti i funzionari del consolato d'Italia a Gerusalemme e tutto il personale diplomatico che è all'aeroporto Ben Gurion nel *desk* informativo (non sono tanti i Paesi che hanno un *desk* informativo all'aeroporto) per cercare di dare consigli ai nostri concittadini. Sono tre giorni e tre notti che non dormono, quindi sono donne e uomini che stanno facendo egregiamente il loro dovere. non abbiamo i numeri esatti delle presenze perché moltissimi non si erano registrati sull'*app* Viaggiare sicuri del Ministero degli esteri e non avevano non avevano l'*app* di geolocalizzazione sempre del Ministero degli esteri. Quelli che l'avevano erano circa 500 e sono stati informati immediatamente attraverso messaggi con un costante contatto. Gli altri si sono materializzati man mano, ad esempio ieri sera un gruppo di 80 persone della Puglia si è fatto vivo con le nostre rappresentanze e sono stati comunque tutti assistiti nel modo migliore possibile, tenendo conto delle difficoltà. Nessuno è stato lasciato solo. Qualcuno può essersi lamentato perché al telefono non rispondevano subito, ma le linee erano intasate perché erano davvero tante le persone che chiedevano aiuto in quella situazione

sono circa un migliaio quelli che abbiamo individuato; 200 sono rientrati questa mattina con due voli militari che la Farnesina ha organizzato insieme al Ministero della difesa; 180 sono rientrati con un volo di una compagnia privata, che ha organizzato sempre il Ministero degli esteri a prezzi molto vantaggiosi. Domani dovrebbero essere imbarcate altre 500 persone con due voli militari e due voli della società Neos. In più, sono

per il giusto verso, tra domani sera e dopodomani mattina non dovrebbero rimanere molti italiani ancora in Israele, Israele, a parte i residenti e coloro che non vogliono partire ovviamente. Comunque faremo tutto il possibile per continuare ad assisterli con grande efficienza ed efficacia, in una situazione che è sempre complicata, anche perché - come sapete - anche in queste ore si sta combattendo nel Nord di Israele. Israele ha evacuato una parte della popolazione al confine con il Libano, Hezbollah sta compiendo attacchi; vedremo se saranno soltanto attacchi dimostrativi per manifestare solidarietà ad Hamas, oppure se sono prodromici di Per adesso non è chiaro, la situazione è sotto monitoraggio, i nostri 1.100 militari

sabato, a livello dei Ministri degli esteri; oltre al Ministro degli esteri di Israele, ho avuto colloqui con il Ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, con il Ministro degli esteri dell'Algeria, con il Ministro

ai quali ho detto che l'Italia sostiene tutte le iniziative favorevoli alla *de-escalation*. Non vogliamo che il conflitto sia allarghi e faremo di tutto per impedire che il conflitto si allarghi al di là della zona attuale. Certo, questo non può significare la rinuncia di Israele all'autodifesa. Israele non può e non deve essere cancellato dalla carta geografica, come ha sostenuto in passato qualcuno e come sta cercando di fare Hamas, il cui obiettivo politico è impedire che ci sia un dialogo tra Israele e un mondo arabo che vuole vivere in una situazione di stabilità e non di guerra. Anche di questo Anche di questo ho parlato con il Ministro degli esteri dell'Arabia Saudita. Quindi, l'Italia sta svolgendo in questo momento anche un ruolo da protagonista. Vi ho detto dell'incontro di domani mattina con il *leader* della Lega araba, ma dovrei incontrare anche il Ministro degli esteri algerino al Cairo e naturalmente i vertici dello Stato egiziano. Per quanto riguarda invece il passato, devo dire che questo Governo non ha mai dimenticato la crisi israelo-palestinese. Una delle mie prime missioni da Ministro degli esteri è stata in Israele e in Palestina; ho incontrato sia il Governo israeliano, sia l'Autorità palestinese; ho più volte incontrato i due Ministri degli esteri. Anche a Roma, come è stato poi riconosciuto in una intervista sul «Corriere della Sera» dal Ministro degli esteri palestinese, l'Italia ha svolto un ruolo proattivo per cercare di rafforzare il dialogo tra le due parti, perché il nostro obiettivo rimane sempre quello dei due popoli e due Stati. Non si pensi quindi che si possa cancellare lo Stato di Israele, che rappresenta una grande democrazia e che non può essere certamente messo sotto scacco. scacco. Esprimiamo anche la nostra solidarietà alla comunità ebraica italiana. Il Governo, come vi è stato già detto più volte, è è impegnato a garantire la sicurezza non soltanto delle istituzioni o delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Israele, ma anche dei luoghi di culto e di riunione dei cittadini italiani di religione Quindi massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti questi nostri compatrioti. Questo è quello che stiamo facendo in sintesi, quindi certamente dialogo e confronto con l'Europa, presenza e contatti e contatti con tutti i Paesi del mondo arabo, oltre che con Israele, che possono essere portatori di pace e di stabilità, che possono favorire corridoi umanitari per la liberazione - ripeto - di donne, bambini e anziani che sono prigionieri nella striscia di Gaza. Gaza. Non vogliamo certamente che si interrompa quel dialogo con il mondo arabo, che ha dimostrato moderazione e che in gran parte coloro che hanno firmato o che erano pronti a firmare gli accordi di Abramo, perché la stabilità e la pace sono il nostro principale obiettivo. Rispondo anche all'appello di chi dice che bisogna avere coesione in politica estera. Mi pare che, in occasione del voto di poco fa alla Camera, si sia dimostrata coesione tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, perché l'opposizione ha votato il testo della maggioranza e la maggioranza votato il testo dell'opposizione. Signor Presidente, concludo esprimendo il parere del Governo sulle differenti mozioni. Sulla mozione presentata dai senatori

che il Governo non condivide. Per il resto, ripeto, a parte il punto 5 della premessa, esprimo parere favorevole. sarà possibile fare una votazione per parti separate, il Governo darà parere favorevole a quel testo. Il Governo esprime parere favorevole anche sul testo proposto dai senatori Borghi Gelmini, Paita.

in questi giorni in Israele, perché la propaganda strisciante - come ha detto il Ministro - sta facendosi spazio. Non vi è in corso - come qualcuno colpevolmente vuol far credere - una guerra tra gli ebrei e gli arabi, tra Israele e la Palestina. Uno Stato sovrano è stato invaso e violentato da una forza terroristica, che, proprio in virtù della sua natura terroristica, esattamente come l'Isis (o Daesch, per i più forbiti), ha preso incivilmente di mira centinaia di migliaia di civili innocenti e inermi. Una forza terroristica è quella di Hamas, che rischia la saldatura saldatura con quella di matrice libanese, gli Hezbollah, in un accerchiamento infernale per Israele; una forza che non possiamo sottrarci dal definire formazione neonazista, in quanto nello statuto stesso di Hamas vi è la cancellazione non dello Stato di Israele, ma dell'intero popolo ebraico. E questo dovrebbero sapere anche i nostri giovinastri dell'Antifa. Personalmente, sono da sempre convinta della necessità dei due popoli e due Stati. Questa carneficina mira proprio ad arrestare quel processo, scagliandosi, oltre che contro gli Accordi di Abramo, contro gli interessi dei tanti palestinesi che, infatti, in queste ore si affastellano alle frontiere, orfani della mediazione dell'OLP e che non si riconoscono in Hamas. Come non si può non parlare di vile neonazismo, che speravamo consegnato alla storia, innanzi alle immagini, che abbiamo ricevuto tutti, noi colleghi, di bimbi di pochi mesi o anni rinchiusi in gabbiette per animali o sgozzati, come nel *kibbutz* di Kfar Aza, nel nord di Israele, dove in realtà nessuno rivendicava quelle terre: è notizia di pochi minuti fa. Come si può non condannare gli avvenimenti e non supportare Israele in una reazione volta a sconfiggere e annientare, giustamente, un terrorismo che ha in mente di espandere la sua influenza, i suoi mezzi e le sue atrocità a tutto il mondo islamico, anche in Occidente?

che nessuno ha deplorato o tentato di arginare; così come il bullismo espresso dai bimbi palestinesi nei confronti del bimbo israeliano catturato da Hamas. L'Occidente ha paura per via del relativismo culturale che ci attanaglia e che rafforza i disvalori del terrorismo di matrice islamica, che nella nostra mancanza di coraggio, di ideali, di orgoglio per la storia trova un varco difficilmente sbarrabile e attecchisce in comunità che già ci circondano e che volutamente non Nell'assunto che la libertà dell'Occidente si difende sotto il muro di Gerusalemme noi dobbiamo crederci. E non bastano mozioni, parole di condanna, cospargersi il capo di cenere, senza memoria: servono fatti solenni. Devono parlare non le armi, ma le coscienze e le idee, che sono sempre state la forza della nostra civiltà. Ecco perché chiederò al presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Alberto Balboni - come già annunciato - di calendarizzare il mio disegno di legge per l'introduzione delle radici giudaico cristiane in Costituzione, confidando che lo facciano anche gli altri Stati europei. Combattere l'indifferenza, come eredi di coloro che stanno subendo gli abomini di questo nuovo olocausto, è la nostra battaglia campale. È infatti nell'indifferenza, cui troppo spesso la nostra società cede, che l'odio trova il terreno fertile per germogliare. Troppo spesso sentiamo ancora predicare l'antisemitismo, la cancellazione di Israele, che - è bene ricordarlo - rappresenta un baluardo di democrazia e libertà imprescindibile, che ha dato una casa a coloro che hanno pagato il prezzo più assurdo e più alto dell'olocausto. Non importa quanto sia buio il presente: si può sempre illuminare il futuro. Questo è il nostro dovere, per onorare le tante piccole Anna Frank di questi giorni, trucidate o costrette a nascondersi in rifugi e tunnel, per sfuggire alla follia generata dall'odio che solamente poco più di settanta anni fa ha travolto l'Europa e il mondo intero, sconvolgendo una generazione intera e che ora si tenta di riproporre con gli stessi metodi crudeli e feroci. L'ingegneria costituzionale non crea né ricostruisce autentici legami sociali. Occorre riannodare il tessuto culturale e sociale brutalmente lacerato dai totalitarismi politici del Novecento e oggi nuovamente minacciati da nuovi totalitarismi religiosi.

invita, in particolare, a tagliare i finanziamenti a tutte le organizzazioni terroristiche, in particolare ad Hamas, protagonista di una drammatica ulteriore deplorevole pagina dell'umanità, confidando sempre nella via diplomatica e nell'aiuto delle comunità musulmane moderate.

Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, membri del Governo, oltre alle tante terribili immagini che inondando il *web* sull'aggressione di Hamas a Israele, ce n'è un'altra che rimbalza spesso in queste ore sulla rete: quella della stretta di meno tra Rabin e Arafat alla presenza di Bill Clinton, trent'anni fa, in occasione degli Accordi di Oslo. speranza, una speranza straordinaria, che oggi appare di molto affievolita, anzi probabilmente affievolita per sempre: la possibilità di una pacifica convivenza tra due popoli e due Stati, lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina. Non dobbiamo essere ipocriti, Presidente: si poteva e si doveva fare di più e meglio, negli ultimi trent'anni, per evitare che i palestinesi venissero segregati in campi invivibili nel Libano. Ho avuto occasione di visitarli e vi garantisco che sono paragonabili alle *favelas* del Brasile. È evidente che, quando giovani generazioni crescono in condizioni disumane, covano al loro interno slanci terroristici che prima o poi esplodono. E questa volta sono esplosi. Quel mondo di Oslo non esiste più, dunque: esiste di nuovo un mondo di violenze, di odi e di estremismi; ed estremismi che non solo si fanno scudo dei destini dei popoli, ma che li piegano e li violentano in nome del loro disegno criminale. Non c'è infatti altro modo per definire il brutale atto di guerra scatenato da Hamas nei confronti di Israele; una guerra che, fin dalle prime battute, si è macchiata di numerosi crimini, in spregio al principio di umanità: rapimenti, esecuzioni di civili, sgozzamento di bambini e di neonati, una strage di giovani nel deserto. Ancora una volta Hamas ha svelato il suo vero volto: attaccare proprio nei giorni in cui il fragile negoziato tra Arabia Saudita e Israele era chiamato a fare dei passi in avanti e farlo con una violenza tale da costringere Israele alla reazione più violenta possibile, a conferma del fatto che a Hamas non interessa affatto la causa palestinese, degli abitanti della striscia di Gaza, ma interessa solo l'eliminazione fisica dello Stato di Israele. E allora, Presidente, per quanto difficile e complicato appaia in questo momento, serve che la comunità internazionale si attivi per scongiurare una spirale di violenza che porterà soltanto a ulteriore odio, lutto e devastazione. Serve coinvolgere - come già si sta cercando di fare - i Paesi arabi moderati, ma anche tutto il resto del mondo possibile, per isolare Hamas e le altre organizzazioni che vogliono cancellare dalla mappa del mondo lo Stato di Israele. Serve anche evitare che la reazione israeliana sia di una furia così cieca e priva del dovuto rispetto per la vita umana da non tenere conto delle ripercussioni future. Bisogna tutelare i civili della striscia di Gaza e tutelare il popolo palestinese, evitando iniziative come quella del blocco dei viveri e dei soccorsi medici. L'Italia e soprattutto l'Europa facciano la loro parte, a cominciare dal delicato lavoro per la liberazione degli ostaggi. Ma, soprattutto, Italia ed Europa tornino a giocare nuovamente un ruolo attivo per tornare un domani all'idea dei due popoli e due Stati e - perché no? - a realizzarla finalmente. Per quanto oggi questa possa apparire una chimera, non ci sono alternative. Non ci possiamo rassegnare al peggio. Grazie, Ministro. Grazie, Presidente.

debba esserci davvero alcun imbarazzo e alcuna reticenza nel definire quello che è stato compiuto da Hamas sabato scorso come un vero e proprio crimine contro l'umanità. La mia condanna, la nostra condanna è nettissima.

un atto infame e vile, che ha preso di mira innanzitutto civili inermi, uomini e donne indifesi, ragazze e ragazzi, bambine addirittura, ammazzati, sequestrati, esibiti come macabri trofei, spogliati, umiliati e privati della dignità. La nostra condanna è totale e crediamo che questo giudizio debba essere condiviso da tutti, istituzioni e società civile, anche ovviamente nel nostro Paese. Gli attacchi colpiscono il popolo israeliano, cui va la nostra solidarietà, e colpiscono anche le speranze del popolo palestinese di veder riconosciuto il proprio diritto alla autodeterminazione, purtroppo tradito sistematicamente negli anni che abbiamo alle spalle. Credo, Ministro, che anche adesso, in questi minuti e in questi momenti, in quelli che sono probabilmente i frangenti in assoluto più difficili di questa lunga e spesso drammatica storia, la politica debba provare ad indicare una strada differente da quella della violenza e della guerra. È per questo che esprimiamo un allarme molto forte per l'*escalation* militare che si sta sviluppando nella striscia di Gaza e che, in aggiunta ai bombardamenti, che peraltro già ci sono stati, rischia di far pagare ad altri civili incolpevoli, quelli di Gaza, un prezzo inaccettabile; civili che peraltro - come lei sa benissimo - non possono nemmeno scappare da quella che è a tutti gli effetti una prigione a cielo aperto perché i valichi - come sappiamo - sono chiusi. È per questo che crediamo che il legittimo diritto alla difesa dello Stato di Israele debba svilupparsi dentro i limiti del diritto internazionale. Ed è per questo che consideriamo gravissimo e inaccettabile che si impedisca alla popolazione civile di Gaza l'accesso a beni essenziali e vitali come il cibo, l'acqua o l'elettricità. Credo inoltre che anche in queste ore così drammatiche dobbiamo cercare di fare tutti uno sforzo per comprendere realmente quello che sta accadendo e anche indagare i motivi - come è stato detto in quest'Aula - per provare almeno a rimuovere gli ostacoli.

il processo di pace sembrava davvero a portata di mano. Ricordo, proprio in quei mesi, un romanzo straordinario del grande scrittore israeliano Abraham Yehoshua, che raccontava il fermento, anche culturale,

dura, erano lontane anni luce dal fondamentalismo e dall'islamismo. E allora io mi faccio e faccio a tutti quanti noi una domanda: come è potuto succedere? Come è stato possibile? Perché l'islamismo, anche in un posto così laico, come era la Palestina, è diventato nel corso del tempo un punto di riferimento addirittura per milioni di persone? Probabilmente, Ministro, questo è successo perché i palestinesi o una larga parte del popolo palestinese si sono sentiti completamente traditi dal mondo occidentale. La *leadership* palestinese che all'epoca si spese per il negoziato, prima e durante gli Accordi di Oslo, è stata con il tempo totalmente delegittimata. Eppure, era una *leadership* laica, che oggi sarebbe utile, anzi utilissima. Lo stesso discorso dei "due popoli, due Stati" è diventato con il tempo una pura finzione e questo mentre la comunità internazionale si girava totalmente dall'altra parte. L'abbiamo denunciato tante volte, spesso in solitudine. Non credo - in - in conclusione - che esistano altre strade: o ci si rassegna a una guerra, un'altra drammatica guerra, peraltro assieme a quella che già insanguina l'Ucraina, una guerra anche in questo caso potenzialmente mondiale, con il rischio concreto della discesa in campo di altri attori; oppure l'Europa cerca di intraprendere un'altra strada. Penso però che, per farlo, occorra restituire verità al tema dei due Stati, provando a garantire i diritti di tutti, la sicurezza di Israele e la protezione del popolo palestinese. Signor Presidente, signor Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la relazione del Ministro degli affari esteri è stata molto puntuale, soffermandosi anche su alcuni dettagli logistici dei quali lo ringraziamo, come pure ringraziamo tutte le donne e gli uomini della Farnesina e dell'unità di crisi. Mi permetterà, signor Presidente, di aggiungere alcuni elementi politici che non ho il tempo di approfondire,

non si parla più di Afghanistan, nemmeno dopo i terremoti con migliaia di morti. Si può discutere quanto si vuole del ruolo dell'Iran: è lì la questione, perché la rivendicazione del ruolo dell'Iran è evidente. che non porterà a un conflitto diretto, ma sicuramente deve portare la comunità internazionale a riflettere su che tipo di postura avere nei confronti di Teheran. C'è un tema: perché ora Hamas, con l'aiuto di Ezbollah e degli iraniani, ha deciso di intervenire? Perché adesso l'Arabia Saudita stava arrivando alla pace di Abramo e sarebbe stato un gesto enorme, che arriverà comunque. comunque. Il momento dell'intervento, però, non a caso è stato adesso. C'è un tema che riguarda i *leader* riformisti arabi, che vanno sostenuti, perché le immagini che a noi fanno ribrezzo, orrore e compassione nel mondo arabo diventano benzina sul fuoco degli estremisti. C'è un tema che riguarda i nostri amici di Israele, e mi limito alla parte politica. Israele è una grande democrazia, che ha mostrato una debolezza: negli ultimi due anni - diciamolo il logorio interno della vita democratica israeliana legato all'instabilità della politica per la mancanza di riforme e alle polemiche sulla riforma della giustizia ha prodotto un indebolimento del sistema israeliano, e chi lo nega nega la verità. Naturalmente, c'è poi un tema di fragilità europea: signor Ministro, non ci siamo. La politica estera europea è del tutto insufficiente e diciamolo che la NATO non basta e che l'esercito comune europeo è, deve essere e sarà un obiettivo di questo Paese. Questi sono soltanto alcuni dei punti politici che avrei voluto affrontare, ma non lo posso fare, per un motivo molto semplice: perché quando a Kfar Azza, un *kibbutz*, 40 bambini vengono decapitati, il dibattito politico viene in secondo piano; perché quando a Be'eri, un *kibbutz*, cento persone vengono sterminate, il dibattito politico passa in secondo piano; perché quando al Nova Music Festival

che non c'è alcun dubbio sulla matrice terroristica dell'attentato di Hamas, ma anche che non c'è nemmeno alcuna possibilità di equiparare Hamas alla reazione controffensiva del Governo democratico di Israele. Chi su questo non dice parole chiare tradisce la causa palestinese. Chi di noi ha detto "due popoli, due Stati" per una vita e lo ha detto non qui, ma di fronte allo Knesset,

per ricordare le parole di un grande premio Nobel per la pace. Oggi parlare di premio Nobel per la pace sembra impossibile, signor Presidente, perché sappiamo che nelle prossime ore la controffensiva sarà violenta.

«Noi vi potremmo un giorno perdonare per aver ucciso i nostri figli, ma non vi perdoneremo mai per averci costretto a uccidere i vostri figli». È qui che sta la grandezza e il dramma

non ci sono parole per commentare quanto sta accadendo in Medio Oriente. La condanna per l'attacco che ha causato allo stato oltre un migliaio di morti e decine di migliaia di feriti non può che essere forte e unanime. È un atto di guerra violento, gravissimo, abominevole. È l'ennesimo episodio di sangue destinato a cambiare la stessa natura del conflitto israelo-palestinese, una questione che da decenni infiamma il Medio Oriente e fa strage di vite umane, donne, bambini, civili innocenti. Non è assurdo dire che con tutta probabilità è per Israele uno dei momenti più tristi e difficili della sua storia recente, un momento di dolore e di rabbia a cui si aggiunge l'apprensione per i tanti ostaggi che mi auguro possano essere presto liberati e possano ritrovare la via di casa. È un nostro dovere, non solo morale, impegnarci e spenderci anche in tal senso. Questo attacco per alcuni versi mi ha riportato alla mente l'uccisione per mano di un estremista di Yitzhak Rabin, un uomo di pace, un simbolo di quel processo di pace israelo-palestinese che non ha mai trovato un punto di arrivo, anche quando un approdo sembrava così vicino e possibile. A distanza di anni la barbarie continua a prevalere sulla ragione e oggi come allora, seppur in modi e contesti molto differenti, la violenza è utilizzata per fermare le evoluzioni possibili, ma il terrore genera solo altro terrore, è destinato a non portare nulla se non dolore, morte e sofferenza. È proprio nel momento in cui i terroristi sembrano ancora una volta avere la meglio che dobbiamo avere la forza e il coraggio di parlare di pace, di pace, di indicare e lavorare per una prospettiva che sappiamo oggi essere necessaria, anche se difficile. Ma questo è il nostro dovere, il nostro compito, il nostro obiettivo. Ogni nostra scelta, ogni nostro atto è e deve essere finalizzato a una simile prospettiva. È quindi proprio nell'ora più buia che tutta la comunità internazionale, nella chiara e ferma condanna di ogni vile e meschino atto terroristico, deve giocare un ruolo attivo. Bisogna farlo sia per impedire che Stati canaglia possano agire indisturbati per sostenere e alimentare più o meno indirettamente i *network* del terrore, sia per evitare - e lo dico con la paura negli occhi - che il truce attentato di Hamas abbia un effetto innesco nella regione e dia la stura a uno o più conflitti di ancor più ampia portata e dalle conseguenze catastrofiche. L'attacco di Hamas in questo frangente non è casuale, è un attacco studiato che ha a che fare più con il futuro che non con il passato, più con la volontà di impedire una normalizzazione, una distensione dei rapporti tra Israele e le principali potenze del mondo arabo che non la ricorrenza dei cinquant'anni dalla guerra dello Yom Kippur. È evidente la volontà di impedire uno sviluppo degli accordi di Abramo che hanno cambiato in meglio la dinamica regionale. Per questo bisogna impedire ad Hamas un successo - mi si passi il termine - politico; bisogna impedire che si blocchi un processo regionale e per farlo bisogna anche affrontare in prospettiva, in una nuova chiave, la questione israelo-palestinese, senza attardarsi in formule più retoriche che nei fatti perseguibili. Le dichiarazioni del ministro Tajani, che ringrazio per la sua continua interlocuzione con il Parlamento, colgono in pieno la delicatezza del momento e contengono l'orizzonte di marcia che la nostra stessa mozione vuole indicare. La necessità di riportare il processo di pace al centro dell'attenzione internazionale, con soluzioni giuste e sostenibili, in linea coi parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza, è un impegno chiaro nella nostra mozione e mi permetto di aggiungere nell'azione del Governo. CRAXI). In conclusione, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia alle due mozioni presentate e condivise con le forze di maggioranza e opposizione, di rivolgere un ringraziamento alle donne e agli uomini dell'unità di crisi della Farnesina, ai nostri diplomatici e al personale di ambasciata che in queste ore stanno lavorando per assicurare il rientro in sicurezza in patria, anche grazie all'impegno dei nostri militari. Al contempo la nostra attenzione e il nostro pensiero vanno ai nostri uomini in divisa, impegnati nella missione United Nations interim force in Lebanon (UNIFIL), che si trovano al confine Nord tra Israele e Libano e sono chiamati a fronteggiare le tensioni che si sviluppano anche su quel fronte. il MoVimento 5 Stelle esprime cordoglio, dolore e sgomento e sgomento per le vittime dell'efferato attacco contro Israele e la sua popolazione civile inerme; un attacco che condanniamo fermamente per la sua brutalità. Esprimiamo anche la nostra più sincera vicinanza ai parenti delle vittime, a quanti in queste ore stanno vivendo l'angoscia per i propri congiunti rapiti dai terroristi. Esprimiamo sgomento altresì, oltre che per la violenza efferata che si è scatenata in un attimo, in una maniera precisa e coordinata sul territorio di Israele, anche per il fatto stesso che questo attacco sia stato effettivamente condotto e portato a termine in uno Stato, quello di Israele, che è noto, che siamo stati abituati a pensare avere una *intelligence* impenetrabile e a confidare nella sua capacità di difesa. In tanti, anche negli interventi che mi hanno preceduto, hanno definito fallimentare proprio quel sistema che avrebbe dovuto sventare e prevenire l'attacco, ma che invece ha dimostrato in maniera inquietante gravissime falle. anche il dovere di sottolineare le responsabilità politiche di un Governo, quello guidato da ormai tempo immemore da Benjamin Netanyahu, che non solo ha abbandonato la strada negoziale, espandendo gli insediamenti illegali, ma ha anche promosso una sistematica politica di segregazione nei confronti dei palestinesi, inseguendo l'ultradestra radicale per bullonare la sua traballante poltrona e, così facendo, ha finito per esporre al pericolo il suo stesso popolo. La comunità internazionale, tutti noi abbiamo osservato questa deriva, ma non è stato mosso un dito per stemperarla, lasciando che la situazione arrivasse al punto in cui siamo.

e incancrenisce; si è smesso di invocare e cercare di perseguire la soluzione che non può che essere quella che anche lei stesso, signor Ministro, ha più volte ricordato ed evocato, ossia quella che il mondo occidentale e il mondo arabo entrambi avevano salutato con favore nell'ormai lontano 1993 e che afferma il diritto a due popoli e due Stati. però vogliamo essere onesti fino in fondo, è necessario collocare questo attacco, questa strage e questa condizione di conflitto in un contesto più ampio, in quella cultura della guerra che si sta pericolosamente diffondendo nell'indifferenza generale, quando non nell'entusiasmo di alcuni; una deriva bellicista e destabilizzante che dall'Ucraina si espande ai confini dell'Europa, dal Baltico alla Moldavia, ai Balcani, al Caucaso al Nord Africa, al Sahel e ovviamente al Medio Oriente. Siamo nel mezzo di quella guerra mondiale a pezzi profetizzata da Papa Francesco, solo che ora quei pezzi rischiano di congiungersi in un drammatico *puzzle*. A questo proposito va detto che non sono confortanti le notizie che arrivano in queste ore da Israele circa la possibile formazione di un Governo di unità nazionale, che al momento - stando alle notizie disponibili - sembra profilarsi con un'impronta ancora più bellicista, ancora più spostato a destra, un esecutivo di guerra: prospettiva, Ministro, che ci auguriamo che il Governo italiano e l'intera comunità internazionale vogliano scongiurare ad ogni costo. Noi ci appelliamo al Governo italiano affinché eserciti ogni azione diplomatica possibile perché Israele eserciti il suo legittimo diritto alla difesa nel rispetto del diritto umanitario internazionale. È urgente altresì l'attivazione di tutti i canali diplomatici per ottenere l'immediata liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. E chiediamo che si lavori affinché da entrambe le parti ci si astenga dal colpire obiettivi civili con azioni indiscriminate, secondo il concetto di punizione collettiva già condannato dall'ONU. Il tempo a mia disposizione sta per scadere. Allora, vorrei chiudere con una notazione politica:

gli sforzi compiuti affinché si potesse avvenire a un testo unico per quanto riguarda quest'Aula sono stati vanificati evidentemente dalla volontà di pochi - neanche di tutta la maggioranza credo - di continuare a utilizzare questa drammatica circostanza in maniera faziosa. Si è finiti, infatti, nella situazione paradossale per cui oggi votiamo tutti favorevolmente i testi di ciascuno

il processo di pace negli ultimi anni è stato messo in grave crisi da iniziative unilaterali da entrambe le parti, come i continui attacchi missilistici provenienti da Gaza e l'allargamento, sostenuto direttamente e indirettamente dal Governo israeliano in carica, degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, cioè una fotografia del reale, fotografia del reale, nonché in linea con quanto da lei affermato poc'anzi. Questo peraltro è quanto gli stessi israeliani, che vogliono la pace, imputano al proprio Governo, ma evidentemente per alcuni pezzi di questa maggioranza questo concetto non è accettabile e non è votabile.

in quanto sotto attacco da parte di estremisti islamici. Vedere giovani aggrediti, rapiti e ammazzati, assistere ai *blitz* nelle case private, dove mamme e bambini sono stati trascinati via come bottino di guerra inorridisce. come inorridisce l'esultazione in nome di Allah, facendo scempio di cadaveri sgozzati ed esibiti come trofei per le vie delle città. Abbiamo visto Noa separata dal fidanzato e portata via in moto dei terroristi, abbiamo visto il suo terrore negli occhi; Shani, seminuda e con le gambe spezzate, caricata sul pick-up degli assalitori che le sputavano addosso;

Di fronte a queste atrocità non possiamo avere tentennamenti nella condanna, che dovrebbe essere univoca, senza se e senza ma. Hamas è un'organizzazione terroristica che ha come obiettivo la cancellazione di Israele. L'attacco di sabato, che ha visto molte vittime tra i civili, è un attacco alla nostra cultura e alla nostra civiltà. Il nostro impegno deve essere orientato ad evitare che vi sia una *escalation*, a favorire un'azione diplomatica che porti ad un cessate il fuoco, alla messa in sicurezza dei civili e alla liberazione degli ostaggi. Se la tensione si allargherà, tutto il mondo sarà in pericolo e il conflitto sarà tra i regimi autoritari e le democrazie occidentali, con il Mediterraneo al centro di un conflitto che porterà instabilità e insicurezza. impegno perché la via diplomatica abbia la meglio deve essere accompagnato dal concentrare l'attenzione su possibili cellule terroristiche nelle nostre città. Non possiamo avere giudici che ritengono che abbiano diritto d'asilo anche terroristi che rischiano trattamenti inumani nei loro Paesi. Chi è terrorista deve essere trattato come tale. Occorre far chiarezza in modo celere sui finanziamenti arrivati anche in Italia da associazioni riconducibili ad Hamas; occorre capire il perché di questi soldi arrivati a queste associazioni, la destinazione, chi ne ha usufruito, la motivazione, perché non è detto che anche nelle nostre città non vi siano delle cellule dormienti; ne va della nostra sicurezza nazionale. Ma per far questo, non possiamo avere uscite fuori dal coro rispetto alla condanna nei confronti di Hamas e l'aggressione nei confronti di Israele. La mozione che tra poco andremo a votare e sulla quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega, ribadisce in particolare la ferma condanna del ricorso a torture e massacri disumani indiscriminati contro la popolazione civile inerme; ribadisce, come già manifestato dal Governo, la piena solidarietà e il sostegno allo Stato di Israele nell'esercizio del suo diritto all'autodifesa; rinnova la condanna più ferma a ogni forma di antisemitismo e impegna il Governo ad agire per evitare che arrivino fondi ad Hamas che vengano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele; a sviluppare un'azione diplomatica con i principali *partner* e attori regionali per evitare l'*escalation* del conflitto. Consentitemi, prima di concludere, che chiederei una preghiera nei confronti di tutte le persone che sono oggi ostaggio di questo gruppo terroristico, e in modo particolare per Doron, Raz,

la condanna all'azione terroristica di Hamas senza se e senza ma. Il motivo per cui il Partito Democratico voterà a favore di tutte le risoluzioni presentate, al di là delle formulazioni e del *wording*, del fatto che potevamo esprimere meglio alcuni concetti o altri. Oggi fa premio il messaggio univoco, affinché tutta la politica dica con chiarezza: no alla violenza *(Applausi)*, no a quelle immagini strazianti che abbiamo visto, con bambini e donne uccise e cadaveri profanati. A cinquant'anni la storia si ripete, anche se non si ripete mai in forme uguali: allora era il 6 ottobre - nel fondamentalismo islamico le date hanno un valore simbolico - e sono tornati a colpire cinquant'anni dopo. Allora erano Egitto e Siria, mentre oggi è Hamas, un'organizzazione terroristica. Penso che da questo punto di vista la risposta deve essere univoca. Noi chiediamo che il Governo si muova, a livello europeo e in tutte le sedi internazionali, per chiedere che le violenze

in generale alcuni Paesi arabi che più hanno rapporti con Hamas hanno un ruolo molto importante per capire se si può aprire una trattativa sulla liberalizzazione degli ostaggi. E questo va fatto, chiaramente, non solo per quelli di origine italiana, ma per tutti. Questo è un nostro dovere. Allo stesso tempo, mi sento di dire, con grande nettezza e forza, che noi abbiamo il dovere, visto che siamo l'Europa, di chiedere che i corridoi umanitari vengano aperti, che il valico di Rafah sia aperto per coloro che vogliono fuggire. Chi conosce Gaza, chi conosce l'urbanizzazione di quei posti, sa che, di quei 2,3 milioni di abitanti, 1,7 milioni sono rifugiati. I ragazzi che hanno che sono quasi un milione, non hanno mai conosciuto un'alternativa a stare dentro Gaza dopo che Sharon l'ha abbandonata al suo destino, nel 2005: persone che sono cresciute nell'odio e nel rancore. Io ho sentito le parole

che hanno subito e subiscono il terrorismo di Hamas. A quelle persone noi dobbiamo dimostrare che l'Europa è diversa. L'Europa non sgozza. L'Europa aiuta chi è in difficoltà. Manda i medici, manda le medicine. *(Applausi)*. Da questo punto di vista, dobbiamo essere uniti, così come dobbiamo essere uniti nel continuare, con perseveranza, ad insistere sul diritto alla pacifica coesistenza di Israele e della Palestina, secondo il modello "due popoli, due Stati". Io sono ben conscio che è complicato e difficile. Non è più come una volta e, a volte, rischia di essere una litania ripetuta per coprire l'impotenza europea. Oggi, però, la comunità internazionale, se non vuole piangere lacrime di coccodrillo, ha il dovere di ripercorrere quella strada. Per poterlo fare, deve sapere che Hamas è intervenuta contro Israele, che è il campo da gioco, mentre carne da macello è la popolazione israeliana e la popolazione civile araba. Lo fa anche per mandare un segnale, neanche tanto cifrato, alle monarchie del Golfo, a coloro che sono antagoniste dell'Islam politico, all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi, a tutti coloro che hanno aperto, attraverso gli accordi di Abramo, una stabilizzazione dell'area che non tiene conto della causa palestinese. Lo hanno fatto in maniera rozza e vergognosa, da condannare. Allo stesso tempo, noi sappiamo che, da questo punto di vista, l'Iran e gli altri Paesi, gli Hezbollah, i

dei "due popoli, due Stati", abbiamo il dovere di condannare con forza, senza se e senza ma, Hamas. Abbiamo bisogno di stare a fianco del popolo israeliano, soprattutto a quello che è sceso portando 500.000 persone in piazza a Tel Aviv, contro un Governo, quello di Netanyahu, che all'interno della sua della sua compagine governativa ha Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Costoro hanno delle responsabilità rispetto ai sollevamenti e alle rivolte avvenute a Jenin. Giocare sul dolore e sulla frustrazione di persone cui viene impedita l'aspirazione al principio di "due popoli, due Stati", che ha a che fare con la possibilità della pacifica coesistenza, vuol dire non riconoscere le difficoltà le difficoltà del conflitto israelo-palestinese. Quindi, se vogliamo bene a Israele, se vogliamo bene a quella democrazia, dobbiamo essere al suo fianco. Dobbiamo stare a fianco di quel popolo e riconoscere che ci sono degli estremisti in quel Governo che non fanno il bene del popolo israeliano.

onorevoli colleghi, non vi nego il momento particolare e vi racconto il perché. Oggi, per me, quest'Aula ha dimostrato l'unione. Ha dimostrato l'unione di intenti. Non cadrò nel tranello di entrare nella polemica, perché non è il momento. È il momento, invece, di raccontare quello che sta accadendo e quello che, a volte, viene addirittura fatto passare come *fake news*, perché le immagini sono talmente aberranti, disumane, barbare. Sabato mattina per il mondo ebraico non era solo lo *shabbat*, ma era una festività che si chiama *Simchat Torah*, che è la gioia della *Torah*. Molti ebrei erano in preghiera nelle sinagoghe; questo avveniva in Italia ed avveniva in altri Paesi del mondo. Quando è arrivata la notizia, i più religiosi avevano addirittura il cellulare spento. E quando è arrivata agli altri, per la paura è passato un brivido dietro la schiena, perché quelle immagini, così violente, si pensava di non doverle vedere più. Uscendo dalla sinagoga quel sabato mattina, sabato scorso, sono inciampata nelle pietre d'inciampo. Le pietre d'inciampo sono quelle pietre che sono state messe lì a testimoniare quello che è accaduto durante le deportazioni e riportano il nome della persona che è stata strappata da quella casa, dalla sua residenza. Lo riportano perché nel *Talmud* c'è scritto che, se si ricorda il nome della persona, si ricorda quello che è stato; se si dimentica il nome, non si può ricordare nemmeno la sua storia. Io pensavo che come quella di andare a prendere le persone casa per casa o di prendere le donne... E guardate che le persone che stavano in quel *rave* non erano di religione ebraica, non erano tutti israeliani: c'erano canadesi, americani, tedeschi, brasiliani. Erano lì a festeggiare e tutti quei ragazzi non immaginavano quello che gli sarebbe successo. Una di quelle ragazze aveva postato qualche giorno prima su Facebook una foto, dicendo "quanto è bella la vita, quanto è bello stare qui a Tel Aviv, la vita è una benedizione". E non ha più fatto ritorno a casa. In un *kibbutz* vicino Gaza vive un ragazzo con cui ho fatto le scuole; sono venticinque anni che adesso vive in quel *kibbutz*. L'ho chiamato, perché ero preoccupata, e mi ha raccontato la sua storia. Vi do il suo nome e il suo cognome, si chiama Daniel Lanternari, così chi ci ascolta può verificare quello che è successo. È stato nel *bunker* con la sua famiglia per tante e tante ore e hanno avuto paura, perché i miliziani entravano nelle loro case. A un certo momento hanno visto uno spiraglio di luce in quel *bunker* e hanno detto "ci siamo, ci stanno venendo a prendere, ce l'hanno fatta". Il Signore ha voluto che si salvassero, ma Daniel - l'ho sentito poco fa per sentire come stava - mi ha detto: «io adesso non so come spiegare poi a mio figlio che il suo compagno di banco non è stato così fortunato, perché è stato preso, non so come spiegare a mio figlio che il suo allenatore di calcio non ce l'ha fatta, perché è stato preso». Questo per dire che quello che è successo sabato è un attentato terroristico, è un attentato alla collettività, è un attentato contro la libertà. Io voglio ringraziare innanzitutto il Governo, e non lo faccio perché faccio parte di un partito di maggioranza, signor Presidente. Lo faccio perché so quello che stanno facendo i funzionari, so quello che sta facendo il Presidente del Consiglio, so quello che sta facendo il Ministro degli esteri per riportare a casa gli italiani, che magari erano lì in vacanza, che magari erano lì in pellegrinaggio, che magari erano lì soltanto per seguire il programma Erasmus, Io dico che bisogna chiamare le cose con il loro nome: questa è una guerra di civiltà, è una guerra di sterminio. *(Applausi)*. Concludo dicendo che quello che sta avvenendo

per cercare di capire le cause, di capire che Israele in questo momento non vuole una guerra di sangue, ma vuole difendersi dal sangue, che è un'altra cosa. Io credo che le mozioni che sono state presentate esprimano al meglio il sentire della nostra Nazione e ringrazio di nuovo il Governo, perché portando qui le persone con quei voli, Ministro, lei sta salvando delle vite e io davvero le sono grata.

la senatrice Mieli per il suo intervento. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

di Hamas contro Israele. Ringrazio i senatori per il senso di comune interpretazione di questa tragedia.